finestra"). Comunico all'Assemblea che in data 11 maggio 2007 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri:* «Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti» "Il link apre una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 31 maggio. Oggi pomeriggio resta confermata la discussione del disegno di legge per l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali. Domani mattina, in apertura di seduta, sarà effettuata la chiama per la votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale potrà indicare tre nominativi per i componenti effettivi e tre per i supplenti. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 12,30. Risulteranno eletti i senatori che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Esaurita la chiama, sempre domani mattina inizierà la discussione del decreto-legge sul ripiano dei disavanzi sanitari, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. A conclusione delle votazioni sul decreto-legge si passerà all'esame del disegno di legge in materia di cognomi della famiglia per la sola discussione generale. La seduta pomeridiana di domani, su richiesta del Presidente della Commissione di vigilanza RAI, avrà inizio alle ore 17 (per concomitante riunione della Commissione) e potrà protrarsi anche oltre il consueto orario. Giovedì 17 maggio, alle ore 10, avrà luogo la riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Gli onorevoli senatori voteranno per primi. Coloro che, per inderogabili esigenze, dovessero chiedere di anticipare il proprio turno nella chiama, sono invitati a farlo con congruo anticipo. Resta confermata nel pomeriggio di giovedì la seduta di sindacato ispettivo. Dopo la tornata elettorale amministrativa, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 29 maggio per il seguito del disegno di legge sui cognomi e per l'esame di ratifiche di accordi internazionali, del disegno di legge in materia di liberalizzazione dell'energia elettrica e del gas, nonché - ove concluso dalla Commissione - della delega sulla sicurezza nei posti di lavoro. In ogni caso, la Conferenza dei Capigruppo è convocata nella stessa giornata di martedì 29, alle ore 12.

su iniziativa del professore Moffa e nell'ambito di un *master* intitolato ad Enrico Mattei, è stato invitato

Robert Faurisson. Si tratta dell'iniziatore del negazionismo, dell'uomo che ha negato l'esistenza delle camere a gas e che si batte per dimostrare che la Shoah è un complotto ebraico.

Faurisson non è uno storico, ma un improvvisato inventore del negazionismo; prima di essere espulso dall'Università di Lione, per questa ragione, insegnava letteratura francese. La lettera con la quale 30 storici italiani hanno protestato e chiesto che l'incontro non avesse luogo è stata definita dall'organizzatore un nuovo documento della *lobby* ebraica. A questo punto siamo arrivati. Credo che la preoccupazione per un evento del genere sia davvero una delle rare cose che possiamo capire e condividere. Non che non debba esservi la libertà accademica di fare quel che si vuole, non che noi vorremmo che a qualcuno fosse impedito di parlare, ma è indecente e indecoroso che un incontro del genere venga organizzato senza che vi sia un contraddittorio, senza che vengano richieste delle documentazioni o delle prove, senza che vi sia un *background* scientifico, senza che la persona appartenga al mondo universitario e tutto ciò, in quanto

- sdegno e preoccupazione molto alta per un episodio di antisemitismo così netto, così grande, così preoccupante nel nostro Paese. Vorrei far notare che l'evento

tende ad attuare in Italia le squadre investigative sovranazionali per rendere più efficiente

che si è manifestato, in maniera virulenta, l'11 settembre del 2001 e che è ancora molto più pericoloso dopo la guerra in Iraq. L'esigenza di rendere molto più efficiente la lotta alla criminalità organizzata transnazionale è stata sentita, per la prima volta, dopo che nel giugno 1985 è stato approvato il Trattato di Schengen, in Europa, che consentiva - anche se in modo graduale - la libera circolazione degli uomini e delle merci all'interno della Comunità Europea senza più controlli alla frontiera.

uno spazio giudiziario comune, cioè ad una collaborazione diretta tra le autorità dei singoli Stati. Come è noto, con i trattati internazionali di collaborazione in materia giudiziaria penale si doveva sempre trattare di una collaborazione tra Stati: la trafila era che l'autorità giudiziaria che doveva ottenere

Tutto ciò comportava una perdita di tempo che rendeva molto spesso inutile la collaborazione giudiziaria penale internazionale, per cui si eliminò questa trafila e si cercò di creare uno spazio giudiziario comune che ponesse immediatamente in contatto le autorità giudiziarie dei due Stati che dovevano collaborare. Il primo accenno a questa esigenza avvenne, in sede di Unione Europea, nel Consiglio di Tampere, dove la Presidenza raccomandò di rafforzare le posizioni dell'Europol, cioè della polizia internazionale europea, attraverso appunto la creazione di squadre investigative comuni che potessero collaborare alla lotta contro le organizzazioni criminali che operavano in via trasversale e transnazionale.

Credo si alluda alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, all'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003 e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003. Al di là di queste considerazioni, è chiaro che si è presentata in maniera più esasperata l'esigenza di collaborazione immediata, effettiva ed efficace

ha favorito - e non poteva non farlo - alcune organizzazioni criminali che hanno stabilito rapporti immediati e diretti con le organizzazioni criminali operanti in Italia.

Come è noto, l'articolo 371-*bis* ha introdotto la Procura nazionale antimafia proprio per la lotta al crimine organizzato in Italia e, in particolare, alle associazioni mafiose. Quindi,

l'intenzione di perseguire una lotta efficace alle organizzazioni che si occupano di traffico di droga e di esseri umani, in passato patrimonio esclusivo delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

la particolare complessità di queste indagini e l'esigenza naturalmente di coordinarle. A questo punto la Commissione ha ritenuto di inserire tra i presupposti anche che i reati siano puniti in Italia con una pena non inferiore a quattro anni

ed ha inserito poi, a solo titolo esemplificativo, i reati che sono menzionati chiaramente nella decisione quadro della Comunità europea e nelle convenzioni internazionali, di cui ho parlato prima, e cioè i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta degli esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione, alla pirateria informatica. è stato inserito anche il principio della doppia punibilità sia nello Stato richiedente che nello Stato richiesto, così come era stato fatto, anche se a titolo diverso,

che, trattandosi di indagini collegate che devono essere coordinate, necessariamente si deve trattare dei reati puniti sia in uno Stato che nell'altro, per cui questa espressione,

La squadra investigativa comune che opera nel territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero dell'indagine. Anche

alternativamente anche «dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo», per il semplice fatto che devono essere applicate per l'operatività in Italia le norme del codice di procedura penale italiano e le nostre norme non prevedono che la squadra di polizia giudiziaria sia diretta dall'ufficiale di polizia giudiziaria, ma in via esclusiva dal pubblico ministero. Questa è stata l'unica ragione per cui è stato eliminato il riferimento all'ufficiale di polizia giudiziaria. Del resto, le squadre di polizia giudiziaria, come tutti coloro che hanno pratica di queste cose sanno, sono normalmente dirette da un ufficiale di polizia giudiziaria che poi riferisce al magistrato delegato e quindi riceve l'istruzione che trasmette in via operativa. L'articolo 371-*quater* disciplina, invece, la costituzione passiva delle squadre investigative comuni; per costituzione passiva s'intende la costituzione che avviene su richiesta di uno Stato estero allo Stato italiano; naturalmente, anche in questo caso si deve trattare di uno Stato della Comunità Europea o di uno Stato che ha ad un trattato internazionale che prevede la costituzione di squadre investigative comuni. Nell'articolo

Repubblica, sentito il procuratore generale, il potere che prima era attribuito al Ministro. Questo è avvenuto perché spetta naturalmente all'autorità giudiziaria verificare sia che l'atto non sia vietato dalla legge

decisione del procuratore della Repubblica sia comunicata allo Stato che ha richiesto la costituzione della squadra e contemporaneamente al

seppur per errore, di bloccare la collaborazione in una materia così delicata, quale quella della lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo. L'articolo 371-*quinquies* disciplina il contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune. L'atto deve contenere il titolo di reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra,

le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni; le modalità di partecipazione di questi esperti che sono designati da altri Stati, organizzazioni

In particolare, stabilisce in un massimo di sei mesi i termini di durata dell'indagine, prorogabili fino ad un anno in caso di indagini già di competenza della procura distrettuale. L'articolo 371-*septies* dispone che i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono compiere attività operativa e sono parificati a tutti gli effetti ai nostri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Faccio notare che questa è una disposizione particolarmente pregnante,

L'articolo 371-*octies*, infine, prevede che possa essere richiesto allo Stato estero con cui è stata costituita la squadra «di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra», quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra

stabilisce che le squadre investigative operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione del L'originario testo prevedeva, sempre all'articolo 4, che le squadre investigative sovranazionali potessero essere dirette anche da un ufficiale di polizia giudiziaria. La Commissione, per le ragioni che ho già esposto, ha ritenuto di disporre che tali squadre non possano essere dirette da un ufficiale di polizia giudiziaria al fine di rendere la norma conforme alle disposizioni del nostro codice penale, che - ripeto - attribuiscono questa possibilità solo al pubblico ministero ed in via esclusiva.

Anche qui la Commissione ha ritenuto che il risarcimento di tali danni da parte dello Stato italiano sia limitato ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune comune e ha soppresso la parte riguardante la rinuncia dello Stato a rivalersi nei confronti dello Stato straniero dei danni cagionati dai loro funzionari nel nostro territorio: questo perché in tutti i trattati internazionali si prevede la possibilità di rivalsa e non si vede perché in Italia non dovesse essere prevista. L'articolo 6 del disegno di

chiedo scusa al relatore perché non sono riuscito a seguire ciò che diceva e non certo per responsabilità sua: in parte per l'impianto audio che è pessimo

immagino più o meno cosa abbia detto; ritengo che abbia illustrato il fatto che questo disegno di legge è la necessaria trasposizione di una decisione quadro che è stata presa dal Consiglio europeo giustizia e affari interni nel 2002.

giustizia e sicurezza, e certamente la costituzione di squadre investigative comuni è una necessità che deriva, in maniera automatica, da questa affermazione di principio. Quindi, noi condividiamo nelle sue linee fondamentali questo disegno di legge che - ripeto - è un atto dovuto del Parlamento nei confronti degli impegni presi allora dal Governo Berlusconi,

Il primo punto è che la decisione quadro stabilisce, in maniera chiara ed inequivocabile, che le squadre investigative comuni devono essere comunicate alla cosiddetta autorità competente, che è un termine di scuola che viene usato in Europa perché - questo è un punto evidentemente importante - ci sono degli ordinamenti giudiziari diversi in ciascuno Stato membro per cui

Bene, in questo disegno di legge non viene identificata; si parla in maniera tutt'affatto generale del procuratore, ma il procuratore può essere chiunque: non è possibile sapere *a priori*, soprattutto da parte di uno Stato estero, qual è il procuratore competente in Italia, atteso che noi abbiamo la giurisdizione che vale per ciascuna procura e vale la questione territoriale. questo punto va assolutamente identificato e precisato; non si può non affrontarlo dal punto di vista legislativo: c'è un vuoto. D'altro canto, chiunque sa che spesso nascono dei conflitti di competenza tra procure; pertanto, se non dirimiamo questa questione, verrà fuori una legge che è zoppa; su questo non c'è nulla da fare. La seconda questione, ancora più importante, riguarda il fatto che questa legge è priva di copertura finanziaria.

a carico dello Stato. Nei fatti non è assolutamente così; non è vero perché, per il semplice fatto che vengono costituite queste squadre investigative, viene previsto che ciascun Stato membro paghi i propri funzionari e quindi lo Stato italiano dovrà pagare tutti i funzionari che andranno all'estero per cooperare nelle squadre investigative in caso di richiesta passiva, cioè di richiesta proveniente dall'estero. Ci saranno quindi fatto che non viene minimamente affrontato dalla legge, che anzi se la cava con questa dizione dell'articolo 6, che non è vera nei fatti. non è vera nei fatti. Poteva essere vera fino a qualche tempo fa, visto che le spese di giustizia finivano nel famoso modello 12 e quindi erano spese obbligatorie; non è più così dal 2002, quando sono stati costituiti due precisi capitoli di bilancio (il 1360 e il 1362) la cui capienza, tra l'altro, è stata tagliata in questa finanziaria. finanziaria. Vorrei sapere cosa pensa la Commissione bilancio di questo tema, visto che qui non è prevista alcuna copertura. Vorrei capire come potrà fare il Presidente della Repubblica a firmare una

(le indagini collegate ci sono anche fra procure italiane); abbiamo aperto uno spazio europeo in cui ormai si circola liberamente,

di giudici che devono favorire i contatti fra le autorità giudiziarie dei vari Paesi e che devono agevolare i contatti di collaborazione diretta.

come avveniva prima la collaborazione internazionale?

in fin dei conti, stabilire una relazione diretta tra le autorità giudiziarie: si parla tanto di Europa e si è realizzata già la libera circolazione delle persone e delle merci, ma non si è fatta la stessa cosa in materia giudiziaria. Soprattutto, si vuole rendere più efficace ed immediata la lotta alla criminalità organizzata, che ha approfittato di queste agevolazioni

che questa raccomandazione hanno sempre fatto, andando anche contro la Convenzione dell'ONU che ha stabilito la costituzione di queste squadre con le quali si fa la collaborazione diretta, per ritornare ad un passato che tutti vogliamo, tutti vogliamo, anche con questa legge, superare proprio per rendere più effettiva ed efficace la lotta al crimine organizzato transnazionale. Non credo pertanto si possa Castelli, che non solo ci farebbe fare un salto indietro nel tempo, ma ci farebbe tornare indietro nell'efficacia della lotta alla criminalità organizzata e soprattutto al terrorismo che, come ho messo in evidenza, è diventato particolarmente preoccupante per tutti gli Stati del mondo.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo,

Il problema è - ripeto - attenersi alla lettera della decisione quadro che richiede l'individuazione di un'autorità competente. Per non creare nuove fattispecie, non ho fatto altro che richiamare il testo, peraltro ricordato anche dal relatore, della legge di trasposizione della decisione quadro sul mandato di arresto. Ho chiesto anche al relatore di fare uno sforzo intellettuale e di individuare una qualsiasi altra autorità, della quale c'è necessità altrimenti la legge non sta in piedi, ma vedo che non riesco a farmi capire e purtroppo

Questo provvedimento se ne va nella più totale indifferenza: è stato appena ucciso un fondamento giuridico del diritto internazionale assolutamente centrale, ma questo Parlamento digerisce tutto.

Presidente, colleghi senatori, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame consentirà di dare attuazione ad uno strumento indispensabile per far fronte ai nuovi sviluppi della criminalità transnazionale, strumento previsto (anche se, finora, mai reso operativo) dagli accordi internazionali stretti dall'Italia con l'Unione Europea e da altri accordi come la Convenzione ONU

comuni sovranazionali, fondamentali al potenziamento della cooperazione giudiziaria e di polizia poiché consentono la conduzione e lo svolgimento sinergico di indagini penali

travalicandone ampiamente i confini, crimini quali il terrorismo, il traffico di armi e di droga, la tratta di esseri umani, la criminalità organizzata. Tramite la squadra investigativa comune, costituita attraverso un accordo sottoscritto tra le competenti autorità di ciascuno Stato, le nostre forze di polizia giudiziaria potranno lavorare a stretto contatto con le forze di polizia di un altro Paese dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, nei diversi territori: ciò consentirà di realizzare azioni mirate ed efficaci, sgombre da ostacoli di forma, per la lotta ai suddetti crimini transnazionali. Per queste ragioni, accolgo

è un problema che stiamo affrontando, con qualche difficoltà, da pochissimo tempo. Non vi è dubbio, infatti, che le squadre investigative siano la parte più intima dell'autonomia dello Stato rispetto alla cooperazione internazionale.

quest'ultima nel contesto dei rapporti internazionali, anche bilaterali, pure con altri Stati. Si tratta, in un certo senso, di un frammento di apertura alla globalizzazione molto più che di apertura all'integrazione europea. che quello che stiamo per approvare sia un provvedimento certamente modesto, certamente limitato, ma di grandi prospettive positive. Per queste ragioni, anche l'UDC voterà a favore, sapendo che si tratta di un esperimento importante, al quale finiamo con il dare corso in Italia sulla base di forti sollecitazioni internazionali non soltanto europee. *(Applausi Presidente, noi avremmo votato volentieri a favore di questo provvedimento, ma, così come è scritto, francamente non possiamo. Capisco Capisco che la questione dell'autorità competente possa essere in qualche modo soggettiva, ma c'è il dato oggettivo della copertura finanziaria. Come facciamo a licenziare un provvedimento di questa natura? In In passato, ci siamo soffermati e bloccati su provvedimenti di legge molto più importanti per questioni molto meno gravi di queste. Oggi, invece, approviamo un disegno di legge senza nessuna copertura.

alla cooperazione internazionale, in un'epoca in cui il crimine organizzato è sempre più transnazionale e vede dipanarsi in vari Stati l'attività criminosa, collegata a traffici di particolare gravità, quali il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il traffico di armi. Era indispensabile, tuttavia, che fossero apportate le modifiche da noi proposte in Commissione che riguardano, limitazione ai reati di maggiore gravità, al fine di evitare attività inutilmente dispendiose, ancorché si tratti di indagini collegate, ma, soprattutto, una limitazione alle organizzazioni criminali. Per esse s'intendono, ovviamente, quelle sussumibili nelle fattispecie previste dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, cioè organizzazioni stabilmente operanti e che svolgono attività di natura criminale, anche se variamente qualificate negli altri Stati dell'Unione Europea, dove non sono sempre presenti reati tipici

e l'attribuzione, comunque, al procuratore della Repubblica, e non al Ministro, della possibilità di interdire atti illegittimi richiesti dall'autorità giudiziaria straniera. Dobbiamo considerare, in ogni caso, che ci poniamo all'interno di un panorama molto articolato e complesso, che andrebbe abbondantemente sfoltito. È vero che oggi, attraverso il Trattato di Schengen, c'è un rapporto diretto tra autorità giudiziarie procedenti, senza bisogno del tramite della rappresentanza apicale politica, però, è altrettanto vero che già nel sistema europeo vi sono organismi, come Europol e Eurojust, che dovrebbero presiedere a questa attività di coordinamento, ma che, in realtà, non funzionano, perché limitati fortemente dalla legge istitutiva, dal tipo di regolamento e dai rapporti con le Polizie (da parte di Europol e Eurojust); c'è poi anche la cosiddetta rete nonché i magistrati di collegamento. Allora, se si vuole davvero arrivare ad uno sfoltimento, ad una maggiore rapidità e ad un vero e proprio coordinamento e collegamento delle indagini, in un'epoca in cui, lo ripeto, il crimine è sempre più necessariamente transnazionale per il passaggio dalle fonti di approvvigionamento a quelle fonti di produzione della materia prima illecita, alla fonte di realizzazione del reato, dovremo pensare ad un sistema molto più snello e più rapido.

il disegno di legge del Governo n. 1271 sull'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali costituisce attuazione di una serie di norme di diritto internazionale. Tra queste, particolare rilievo assumono la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 e la decisione quadro del Consiglio d'Europa del 13 giugno 2002. Pur in ritardo nell'ossequio agli obblighi internazionali assunti, l'approvazione del presente disegno di legge viene a riempire un vuoto normativo interno e in concreto dà un supporto legislativo e ordinamentale importante nell'ambito della cooperazione tra Stati, anche in materia di indagini e di investigazioni criminali. Negli ultimi anni abbiamo assistito tutti ad una particolare virulenza della grande criminalità e del terrorismo; di fatto è successo più volte che le barriere giuridiche e istituzionali ancora esistenti tra gli Stati europei abbiano causato rallentamenti e perdite di efficienza nelle indagini della magistratura e della polizia giudiziaria. Da più parti, nazionali e internazionali, si è avvertita la necessità di superare ostacoli formalmente e apparentemente insormontabili. Da più parti si è sollecitato l'intervento anche del Governo e del Parlamento italiani per adeguare la nostra normativa e per dotare le nostre forze di polizia e la magistratura degli strumenti più adeguati nella lotta alla criminalità, di qualunque genere essa sia. Di particolare significato sono alcune delle norme che oggi siamo chiamati ad approvare. Innanzitutto, è comunque fondamentale il richiamo agli accordi e alle convenzioni internazionali nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale. L'esperienza e la prassi investigative ci hanno insegnato da molto tempo come non sia possibile individuare i responsabili dei maggiori fenomeni criminali che hanno ormai certamente una caratura e una valenza internazionali, se non grazie alla collaborazione degli organi di investigazione stranieri; collaborazione che deve essere piena e reciproca. Per questo, riteniamo in maniera convinta che l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali sia una risposta sicuramente valida alle esigenze emerse e prospettate. Il tutto, peraltro, nell'ottica del rispetto delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale: la creazione di queste squadre ad iniziativa dei procuratori della Repubblica, la vigilanza sul rispetto delle norme e delle procedure ad opera del procuratore generale presso la Corte d'Appello, la direzione delle squadre da parte del pubblico ministero delegato alle indagini, la dovuta informazione ai Ministri della giustizia e dell'interno. L'istituzione di queste squadre è prevista nell'ambito delle norme del codice di rito penale vigenti e in presenza di precisi e specifici presupposti accuratamente indicati, tra cui: i motivi per cui si procede alla sua costituzione, gli atti da compiere assieme ai colleghi stranieri, la durata delle indagini stesse, l'utilizzazione del materiale probatorio raccolto. In sede di Commissione giustizia sono state apportate alcune modifiche al disegno di legge del Governo, secondo le specificazioni illustrate dal senatore relatore. Tali modificazioni sono state apportate per meglio adeguare questo nuovo strumento investigativo alle garanzie istituzionali e personali già previste dal nostro codice. Nel passato anche recente, infatti, le indagini più delicate si sono scontrate a volte con l'impossibilità di utilizzare e valorizzare il materiale probatorio individuato *in nuce* dai nostri organi investigativi. L'auspicio, con questa nuova normativa, è quello di superare formalismi e barriere che nell'epoca moderna e soprattutto nell'ambito comunitario non hanno più alcun senso, non hanno più alcun senso, specialmente con gli ultimi allargamenti dell'Unione Europea. Anzi, in tale ottica, proprio l'approvazione del presente disegno di legge consentirà un'efficienza ed un'efficacia maggiori delle nostre forze investigative. L'aumento della libera circolazione delle persone e dei beni a livello continentale ha creato maggiori problemi nella fase di accertamento dei reati; ben venga, quindi, l'accoglimento di una sollecitazione che ci arriva anche dai Paesi esteri. L'Italia persegue ormai da tempo la strada della massima collaborazione a livello internazionale, in ciò concretizzando e attualizzando alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione, convinta che solo la collaborazione internazionale e i pacifici rapporti tra popoli e Stati possono contribuire ad uno sviluppo armonico e più giusto della nostra società.